L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni. Sarà svolta

in risposta all'interpellanza in oggetto, riferisco preliminarmente gli elementi conoscitivi acquisiti dal Ministero dell'interno, utili alla ricostruzione della vicenda. L'Angelo Mai è un ex convitto, sito nel Rione Monti di Roma, abusivamente occupato dal novembre 2004 dal "Comitato popolare lotta per la casa". L'Amministrazione capitolina, dopo avere acquisito l'immobile dall'Agenzia del Demanio, ha comunicato agli occupanti la necessità di ristrutturare l'edificio per adibirlo a plesso scolastico. Nella zona, infatti, vi è carenza di queste strutture e tale situazione è stata più volte lamentata dagli stessi cittadini residenti. Il XII dipartimento del Comune di Roma, competente per materia, ha commissionato i lavori di ristrutturazione dell'immobile e, in attesa della consegna alla ditta appaltatrice, ha intrapreso delle trattative con gli occupanti abusivi per riuscire a rientrare bonariamente nella disponibilità della struttura. Nel luglio 2006 la ditta appaltatrice ha preso possesso dell'edificio, lasciando che gli occupanti continuassero ad occuparne soltanto una porzione e concedendo sessanta giorni di tempo per l'abbandono definitivo. Il 4 ottobre 2007 il personale del Corpo della Polizia municipale-Nucleo pronto intervento centro storico, decorso inutilmente il termine fissato per lo sgombero, si è recato *in loco* per fornire assistenza alle operazioni di delimitazione dell'area di cantiere; una volta delimitata l'area, è stato interdetto l'accesso a tutti gli estranei per ragioni di sicurezza. Inoltre, è stata autorizzata la presenza di dipendenti dell'Ufficio decoro urbano per coadiuvare gli occupanti nelle operazioni di trasloco, permettendo a questi ultimi di accedere nell'edificio nel numero massimo di due per volta, al solo fine di ritirare gli effetti personali. Lo sgombero, quindi, non è stato eseguito in maniera forzosa, poiché non era stato previsto l'intervento della forza pubblica. Secondo quanto riferito dal Nucleo pronto intervento centro storico del Corpo della polizia municipale di Roma, intorno alle ore 10 circa del 4 ottobre 2007, davanti all'ingresso dell'istituto, si è radunato un nutrito numero di manifestanti che ha controllato dall'esterno, in modo pacifico, lo svolgimento delle operazioni. Dopo circa mezz'ora sono sopraggiunti i senatori Bonadonna e Martone il consigliere regionale Giuseppe Mariani, i quali, insieme all'assessore alle politiche sociali del I municipio, Perrotta, già presente dall'inizio delle operazioni, hanno chiesto delucidazioni al personale della polizia municipale su quanto stava accadendo all'interno. In un secondo momento, i parlamentari si sono nuovamente rivolti al personale del Nucleo di pronto intervento, chiedendo di accedere all'interno dell'edificio per verificare le circostanze riferite. Gli agenti della Polizia municipale hanno negato l'accesso per motivi di sicurezza, posto che non erano ancora stati messi a punto gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità delle persone nelle aree di cantiere. Sempre secondo quanto riferito dagli agenti, le personalità predette, pur avuta notizia del rifiuto, hanno ugualmente cercato di oltrepassare il blocco costituito da personale della Polizia municipale e da un'autovettura di servizio, inscenando una protesta nel corso della quale è stata anche danneggiata tale autovettura. Nella circostanza, così come riportato nella nota redatta dalla Polizia municipale, alcuni agenti hanno riportato lesioni personali; anche l'assessore alla Regione Lazio Giuseppe Mariani, in seguito ad una caduta, si è ferito ed è stato soccorso con un'ambulanza. Il procuratore della Repubblica di Roma ha riferito che per i fatti menzionati nell'interrogazione è stato iscritto il procedimento penale n. 42787/ 2006, a carico dei senatori Salvatore Bonadonna e Francesco Martone e di alcuni consiglieri regionali per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali ai danni di agenti della Polizia municipale di Roma. In data 19 gennaio 2007 è stata avanzata richiesta di archiviazione, tuttora pendente dinanzi al GIP. Quanto alla questione del possibile danno determinato dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato, va rilevato che nessun danno può scaturire di per sé dal solo fatto dell'iscrizione, che ha natura di atto segreto, non comunicabile, ai sensi dell'articolo 335, 335, comma 3, del codice di procedura penale, se non ai diretti interessati (indagati, difensori e parti offese) e nei soli casi previsti dalla legge. Un possibile *vulnus* può derivare piuttosto dalla indebita divulgazione delle notizie riservate, ma ciò evidentemente non attiene alla problematica dell'iscrizione, bensì a quella della tutela del segreto delle indagini. Peraltro, in materia di iniziative legislative volte a modificare l'attuale regime normativo dell' iscrizione del nominativo della persona nel registro degli indagati, deve farsi presente che anche questo tema è all'attenzione della commissione di riforma del codice di procedura penale presieduta dal professor Giuseppe Riccio, istituita dal Ministro della giustizia poco dopo il suo insediamento ed i cui lavori saranno conclusi tra breve.

il rapporto degli agenti della Polizia municipale sia del tutto fantasioso; infatti, siamo di fronte ad una richiesta di archiviazione da parte dello stesso magistrato. È del tutto falso. Mi riesce difficile pensare che

di grande momento, signor Sottosegretario, che attiene, come discrimine giuridico, all'articolo 68 della Costituzione.

delle forze dell'ordine. Sta di fatto che gli agenti della Polizia municipale hanno negato a due parlamentari ogni possibilità di ingresso all'interno dei locali del Centro sociale Angelo Mai. Peraltro, mi pare che la manifestazione di protesta per lo sgombero fosse non solo di massa, pacifica e non violenta, ma ma anche fortemente radicata all'interno di un consenso che vi è nel quartiere per un Centro sociale che svolge anche un'attività culturale, educativa e pedagogica di massa

che ben conoscono i limiti della propria azione e ben sanno che le proprie opinioni e le proprie azioni sono coperte dall'articolo 68 della Costituzione soltanto quando sono proiezione, prosecuzione del mandato parlamentare (e quindi sono ben consapevoli di quale sia il discrimine), sono stati non solo bloccati nella loro azione, ma poi hanno ricevuto un rapporto

della tutela delle funzioni, delle garanzie e delle prerogative dei parlamentari. Senza tale tutela, ognuno di noi, nel momento in cui ritenesse, come noi riteniamo, che il ruolo del parlamentare non sia solamente quello di parlare in Aula o di esprimere opinioni

Con l'accordo intergovernativo del 24 novembre 2006 è stato previsto il riprocessamento in Francia del combustibile nucleare irraggiato italiano. La società Sogin, quindi, ha posto in essere le procedure occorrenti per definire gli aspetti contrattuali con l'Areva in vista della stipula finale. Il rinnovo dei vertici della società Sogin spa, avvenuto nei primi mesi dell'anno, non ha influito su tali procedure alle quali, nel corso dei necessari perfezionamenti, ha partecipato anche il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di sua competenza, al fine di valutare la congruità dello stipulando contratto con gli accordi intergovernativi. In data 2 maggio 2007, è stato firmato dal ministro Bersani e dall'omologo francese onorevole Francois Loos un *addendum* all'accordo italo-francese del 24 novembre 2006 per la definizione di alcuni aspetti, in merito ad eventuali problematiche che potrebbero insorgere in fase di applicazione dell'accordo stesso. Il 9 maggio 2007, a seguito della firma del predetto *addendum*, è stato, quindi, concluso il contratto tra la Sogin spa e Areva. Il contratto ha un valore di oltre 250 milioni di euro, implementa i citati accordi intergovernativi e prevede il trasporto, il trattamento e il condizionamento del combustibile irraggiato italiano. L'obiettivo del contratto con l'Areva è quello di avviare le operazioni di trasporto del combustibile già entro il corrente anno, iniziando dalla centrale di Caorso (per il cui combustibile sono previste 16 spedizioni), per proseguire - non appena avuta la disponibilità dell'apposito contenitore - con il trasporto dal deposito di Avogadro dove, al termine delle attuali operazioni di trasferimento del combustibile dalla piscina Eurex, sarà presente combustibile del Garigliano (dal (dal quale sono previsti dieci spedizioni), per finire con i trasferimenti dalla centrale di Trino (da cui sono previste tre spedizioni).

(il narcisismo è di tutti) nei vari articoli di giornali, dove vengono processati, si promettono efficienze incredibili e si dice "l'uomo chiamato dal Tesoro a rivoltare la società Sogin come un calzino dopo gli scandali della passata gestione". Si Si dice che serve più efficienza e più competenza, ma, se *decommissioning* ci dev'essere, si deve fare una scelta politica: ci vuole, cioè, il posto dove portare i rifiuti nucleari. Questo Paese deve dire se vuol mettere i rifiuti nucleari in un posto in alto, in un deposito

qual è il piano industriale delle attività di *decommissioning* perché, al di là delle cose che si possono dire sul giornale, il piano industriale va fatto, ma, se non c'è l'indicazione del sito, è evidente che il *decommissioning* non avverrà. E questa cosa va detta ai sindaci,

della firma dell'accordo dai giornali, mentre prima, con la gestione tanto vituperata da alcuni dall'amministratore delegato, quantomeno c'era stato lo sblocco di alcune situazioni di conflittualità e c'è stato un accordo

al fine di migliorare la concorrenza nel settore dei servizi, l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo risultante dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, dettato apposite disposizioni finalizzate ad accrescere la trasparenza e la libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi Internet. In particolare, in merito all'applicazione della norma relativa all'eliminazione dei costi di ricarica, numerose sono state le segnalazioni pervenute sinora sia da parte di oltre 130 consumatori, che di associazioni di consumatori, inerenti alla modifica unilaterale dei piani tariffari e di singole voci di costo da parte di alcuni operatori di telefonia mobile. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta dal Ministero dello sviluppo economico, tali segnalazioni sono state tempestivamente trasmesse all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in qualità di organo competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 40 del 2007, svolge il compito di vigilare sull'attuazione dell'articolo 1 nella sua interezza e stabilisce le modalità attuative del comma 2 dello stesso articolo, relative alle voci di costo che compongono l'offerta, comminando inoltre le sanzioni in caso di violazione della normativa, al fine di aumentare la trasparenza dei prezzi e rendere facilmente confrontabili le offerte commerciali. Il Ministero, quindi, non è deputato a valutare il comportamento dei singoli operatori - nuove offerte commerciali, variazioni di profili tariffari per cui, ove gli operatori ritengano di compensare il mancato introito per i costi di ricarica, in conseguenza dell'abolizione degli stessi, con profili tariffari che determinano un aumento del costo del servizio, questo deve essere valutato dagli operatori stessi, tenendo conto che in un mercato concorrenziale, com'è noto, il prezzo non è una variabile ininfluente nelle decisioni di acquisto. Compito del Ministero è, bensì, osservare ed analizzare gli effetti complessivi sui consumatori dell'eliminazione dei costi di ricarica e delle altre misure legislative adottate, al fine di aumentare la trasparenza e la concorrenza nei settori della telefonia fissa e mobile. Per quanto riguarda la riduzione dei margini per gli edicolanti e giornalai e, comunque, per i distributori delle ricariche telefoniche, premettendo, secondo anche quanto riferito dal Ministero delle comunicazioni, che all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è affidato, ai sensi della legge n. il compito di regolare le relazioni fra i gestori di telefonia e gli utilizzatori dei servizi nei limiti dell'autonomia contrattuale delle parti, la stessa Autorità, in questo ambito, non dispone di alcun potere di intervento. In merito a tale problematica, il Ministero dello sviluppo economico, temendo disagi per i consumatori derivanti dal possibile conflitto fra gestori di telefonia mobile e distributori, ha convocato le parti il 17 maggio scorso (alla presenza del collega sottosegretario onorevole Bubbico). Nel corso di un primo incontro, presenti i rappresentanti della Federtabacchi e i quattro gestori di telefonia mobile Vodafone, Wind, Tre Italia e Telecom Italia, è stata lamentata da parte della Federtabacchi, soprattutto la riduzione dei margini nella vendita delle ricariche. L'invito caldeggiato dal rappresentante del Governo è stato quello di addivenire ad una soluzione a garanzia del servizio. Le parti hanno assunto l'impegno ad effettuare incontri bilaterali, separatamente tra singoli gestori e la Federazione dei tabaccai, allo scopo di individuare soluzioni innovative e più razionali nel campo della distribuzione che permettano un abbattimento dei costi, senza pregiudizio per i margini dei distributori. Il sottosegretario di Stato ha, altresì, incontrato l'Assotabaccai e l'AGEMOS. Entrambe le associazioni si sono impegnate ad effettuare incontri con le rispettive controparti per l'individuazione di possibili soluzioni, anche sotto il profilo della razionalizzazione della distribuzione, per il conseguimento, in questa fase, di economie. Il Ministero dello sviluppo economico cercherà di favorire, nel rispetto dei differenti ruoli, tutte quelle soluzioni che possono agevolare la definizione di un accordo delle parti, per evitare disservizi e disagi per l'utenza.

guadagno - evidentemente eccessivi - delle grandi compagnie adesso li vogliamo ridurre ai giornalai, ai tabaccai e alle altre rivendite. Dico questo perché a me convince

di più: «Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe (...)»; e, infine, al comma 2 si aggiunge: «L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta (...)», è del tutto evidente che tra queste voci sia incluso anche il costo all'ingrosso per i distributori. Attenzione. Qui c'è un tema più di fondo, che, per quanto riguarda la mia parte politica, noi poniamo: la giusta politica di liberalizzazione, quella che serve ai consumatori, se è una politica tesa a favorire il consumo dei ceti più deboli (cosa fondamentale che, più che del cittadino consumatore, preferiamo parlare del cittadino lavoratore, del cittadino operatore sociale), se serve a permettere l'accesso a beni e servizi a ceti deboli, ovviamente una politica un po' controproducente se noi da una parte dessimo e dall'altra togliessimo. Nello stesso tempo, anche i gestori delle rivendite - penso ai tabaccai, ai giornalai - sono soggetti che avrebbero delle forti difficoltà.

(quello che toglie l'obbligatorietà del costo della ricarica, in un quadro europeo che addirittura vuole togliere i costi per le telefonate a livello europeo),

Grazie, senatore Tecce, perché lei è uno dei pochi che tiene in vita l'istituto delle interrogazioni in questa Camera. La ringrazio anche per questo.

sull'argomento relativo alle difficoltà finanziarie delle istituzioni scolastiche il ministro Fioroni ha riferito alla settima Commissione della Camera nel corso dell'audizione svoltasi il 24 aprile scorso. Come già riferito in quella sede, con le leggi finanziarie del periodo 2002-2006, sono stati tagliati il 72,6 per cento dei fondi per gli esami di Stato, il 46,6 per cento dei fondi per le supplenze brevi e il 53 per cento dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico. Presumibilmente, i tagli sono stati fatti operando su cifre di bilancio ritenute eccedenti rispetto alle esigenze che sono state, quindi, sottostimate. In particolare, per gli esami di Stato, il taglio del 72,6 per cento delle risorse è stato operato ritenendo che, a seguito della normativa allora introdotta sulla composizione delle commissioni esaminatrici, le risorse in precedenza stanziate per tale finalità fossero in eccesso e non tenendo presente, invece, che già mancavano oltre 180 milioni di euro per pagare le commissioni per gli esami di Stato già svolti. Uno dei problemi che il Governo ha dovuto affrontare appena insediato è stato proprio quello di reperire subito le risorse necessarie per assicurare il regolare svolgimento della sessione degli esami di Stato per l'anno scolastico 2005-2006. In un difficile contesto di finanza pubblica, si è provveduto a questa impellente esigenza con il decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, che ha elevato di 63 milioni di euro per l'anno 2006 il limite di spesa stabilito dalla legge n. 448 del 2001. Quanto alle supplenze brevi, il taglio è stato operato non tenendo conto che buona parte del debito già accumulato dalle scuole riguardava proprio le supplenze e, in particolare, le supplenze per maternità. Queste ultime, come è noto, non sono eludibili né razionalizzabili ed hanno nella scuola un'incidenza maggiore rispetto alla media degli altri comparti del pubblico impiego, in considerazione che circa l'80 per cento del personale è di sesso femminile, principalmente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Bisogna poi tenere anche conto della pronuncia della Corte costituzionale in base alla quale la «supplente breve» che entra in maternità è a carico della scuola al 100 per cento. Per queste considerazioni, il ministro Fioroni ha inviato al Ministro dell'economia e delle finanze formale richiesta affinché le spese per le supplenze legate alla maternità di titolari e supplenti non siano poste a carico del bilancio delle scuole. Per quanto concerne, poi, il pagamento della tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani da parte delle istituzioni scolastiche, va preliminarmente ricordato che con l'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sulla base del parere n. 1784 del 1996 del Consiglio di Stato, che considerava l'onere in questione rientrante tra le «spese varie d'ufficio», di cui all'articolo 3 legge n. 23, e su conforme avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'anno 1999 furono emanate, rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno e delle finanze, tre apposite circolari con le quali l'onere in argomento veniva riconosciuto in capo ai Comuni per le scuole dell'obbligo e alle Province per quelle superiori. Successivamente la questione, su iniziativa degli enti locali interessati, fu portata più volte all'attenzione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali con alterne vicende, fino all'ultima decisione assunta nel corso della riunione del 6 settembre 2001, nella quale - anche sulla scorta della sentenza n. 4944 del 9 febbraio 2000 con la quale la Corte di cassazione decideva un contenzioso specifico, avviato nel lontano 1989 cioè, della legge n. 23 del 1996), ponendo l'onere a carico dell'amministrazione scolastica - si assumeva che le spese per la tassa in parola fossero "a carico dello Stato". Contestualmente si affermava la necessità di reperire un apposito stanziamento in bilancio e si rinviava ad un incontro tecnico per la determinazione della cifra annua attribuibile forfetariamente ai Comuni per la tassa in discorso; cifra, questa, successivamente quantificata, d'accordo con gli altri soggetti interessati, in 75 miliardi di lire. A tali fini, i vari decreti, relativi alla ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato, hanno stanziato solo per il primo anno (2002) la somma di 38.734.267 euro (incardinandola, peraltro, impropriamente e "pericolosamente" in un capitolo di bilancio destinato alla "integrazione delle spese di funzionamento"), provvedendo nei successivi esercizi finanziari ad appostare cifre diverse e progressivamente inferiori; il che ha determinato le note conseguenze a seguito della decurtazione del 53 per cento dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, operata senza tener conto che tale voce di bilancio comprende anche la spesa obbligatoria per la TARSU. Per la TARSU si sta lavorando con tutti i soggetti istituzionali cointeressati per trovare un'idonea, possibile soluzione normativa condivisa. È anche stato presentato alla Camera il disegno di legge n. 2272-*ter*, che speriamo il Parlamento possa approvare per una soluzione definitiva di tale spinosa questione.

cioè la finanziaria 2007, pur contenendo misure di razionalizzazione della spesa, che peraltro non incidono sulla qualità e quantità dell'offerta formativa complessiva, reca importanti misure a favore della scuola, per il potenziamento dell'autonomia scolastica, per lo sviluppo e la qualificazione del sistema dell'istruzione e per la valorizzazione del personale scolastico. Per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 601, della suddetta legge, i fondi assegnati alle istituzioni scolastiche, pari ad oltre 3 miliardi di euro, con un valore medio per ogni scuola intorno ai 300.000 euro, sono stati accorpati in due soli grandi capitoli di bilancio (spese per il funzionamento amministrativo e didattico e spese e sono assegnati direttamente dal Ministero alle istituzioni scolastiche. Trattasi di una misura che mira alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, oltre che alla semplificazione e snellimento del procedimento di accreditamento alle scuole. Infatti, l'accorpamento in due soli grandi capitoli del bilancio dello Stato consente alle scuole autonome di definire le priorità di spesa per l'attuazione del loro piano di offerta formativa, senza subire destinazioni vincolate e predefinite, come è invece avvenuto Tale scelta, oltre a rendere più trasparente il processo di finanziamento delle scuole, lo accelera eliminando il passaggio dagli uffici scolastici regionali alle contabilità speciali degli uffici scolastici provinciali e da questi alle scuole. Tornando alle difficoltà finanziarie delle istituzioni scolastiche, è noto che il Ministero, per risolvere le situazioni più critiche e per evitare conseguenze negative sul funzionamento delle scuole, ha dato indicazioni agli uffici scolastici periferici per l'urgente accreditamento alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie già disponibili sulle contabilità speciali; trattasi di somme importanti che, pur non risolvendo per intero le difficoltà, hanno consentito una copertura significativa dei debiti, soprattutto in relazione al mancato pagamento del personale supplente. Il Ministero, inoltre, attraverso monitoraggi svolti dagli uffici scolastici regionali, ha proceduto all'accertamento dell'effettivo fabbisogno delle scuole; sulla base degli esiti di tale accertamento, si provvederà ad erogare una specifica integrazione per le supplenze brevi e per i compensi alle commissioni degli esami di Stato. Con riguardo ai finanziamenti disposti direttamente dal Ministero alle scuole per l'anno 2007, in attuazione della legge finanziaria, sono state già erogate alle istituzioni scolastiche la prima e la seconda quota; la terza sarà esigibile dal 26 giugno prossimo. Per completezza di quadro espositivo, va detto altresì che la dotazione finanziaria assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri e parametri contenuti nel decreto ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007, non esaurisce la totalità delle somme da trasferire alle scuole per l'anno 2007, ma rappresenta soltanto una quota, alla quale devono essere aggiunti: gli importi da determinarsi, autonomamente, dalle scuole, riguardo ad alcuni istituti contrattuali nonché ad altre spese già giuridicamente definite; le integrazioni finanziarie che saranno disposte, a seguito di rilevazione dei dati oggettivi relativi alla gestione dell'anno di riferimento; le assegnazioni finanziarie che continueranno ad essere disposte dagli uffici scolastici regionali e dagli uffici scolastici provinciali; gli ulteriori finanziamenti che saranno disposti, nel corso dell'anno, sulla base di specifiche disposizioni normative, quali quelli relativi al fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa istituito dalla legge n. 440 del 1997, somme aggiuntive da legge finanziaria, e così via. Sono ora allo studio iniziative normative per un'idonea soluzione dei problemi finanziari delle istituzioni scolastiche. Con la legge di assestamento di bilancio si cercherà di dare una prima risposta in tal senso, per risolvere i problemi più urgenti. Con riguardo, poi, a quanto lamentato nell'interrogazione circa l'aggiornamento del *software* fornito alle scuole per la gestione delle attività amministrative, faccio presente che, per aggiornare tempestivamente il pacchetto *software* sulla base delle novità che ogni anno sono presenti nelle leggi finanziarie, la competente Direzione generale del Ministero della pubblica istruzione si rivolge al Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di avere indicazioni corrette e certificate su come aggiornare il pacchetto. Le indicazioni per il 2007 sono arrivate a metà del mese di febbraio, conseguentemente il 12 marzo scorso l'aggiornamento del *software* è stato messo a disposizione delle istituzioni scolastiche. Quanto alla velocità con la quale gli altri produttori di *software* rilasciano i loro aggiornamenti, vorrei fare presente che si ritiene prioritaria, oltre che la tempestività, anche la correttezza e certificazione delle soluzioni che vengono fornite, al fine di evitare ulteriori situazioni di disagio. Grazie.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, devo dire che non sono del tutto soddisfatta della risposta, che comunque è molto articolata e puntuale, ma che forse non coglie il senso delle nostre domande.

si è giustamente inaugurata una nuova modalità di finanziamento delle scuole, con il famoso «capitolone», considerata la lentezza dei tempi per decidere questo tipo di modalità,

a ristrettezze e tagli dal 2002 e quindi soggetto a un lavoro defatigante di resistenza, di autosufficienza e di tenuta determinato dal consumo delle proprie risorse economiche. Tale collasso economico ha determinato una grave situazione di lesione dei diritti: dei supplenti, che non sono stati pagati per mesi; degli studenti, ai quali molte volte non è stata garantita la supplenza per mancata mancata nomina da parte dei dirigenti che non si assumevano la responsabilità di nominare i supplenti. Penso quindi che

come mai - questa è una domanda anche autocritica che si devono porre il Governo e la maggioranza - non ci si è resi conto della situazione delle scuole? La risposta interroga due responsabilità. In primo luogo, quella politica, perché era da mesi

una verifica delle capacità del Ministero, l'organo dello Stato che garantisce la continuità, di cogliere

quanto vada attribuita a precedenti amministrazioni, il Governo deve assumersi fino in fondo. Non sono, inoltre, soddisfatta delle risposte

di un ente che non garantisce l'efficienza e soprattutto fa sì che le scuole molte volte non riescano a connettersi in determinati orari per cui ne rallenta moltissimo il lavoro, obbligando

istruzione*. Signor Presidente, vorrei premettere che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la finanziaria per il 2007) il Governo ha approvato un articolato piano di interventi per il rilancio complessivo del sistema di istruzione; tra i vari interventi è stato previsto un incremento dello 0,4 per cento del valore medio nazionale del rapporto alunni-classe (dalle attuali 20,6 a 21 unità di allievi per classe) al fine di realizzare, nel rispetto della vigente normativa, una più efficace determinazione e distribuzione delle risorse disponibili. La relazione di accompagnamento della legge finanziaria, facendo riferimento al numero degli alunni in base al quale è stato determinato l'organico di diritto dell'anno scolastico 2006-2007 (un docente per 10 alunni), ha stimato in 19.039 i posti da ridurre per raggiungere l'obiettivo prefissato. Questo numero si è ridotto a 11.726 unità anche per effetto dell'introduzione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione e per l'incremento della popolazione scolastica, stimato in oltre 28.000 unità. Di queste 11.726 unità, soltanto 7.053 posti deriveranno dall'intervento di razionalizzazione degli organici di diritto, secondo le tabelle allegate allo schema di decreto interministeriale sugli organici di diritto per l'anno scolastico 2007-2008. Tale numero non incide sulla qualità complessiva del servizio d'istruzione. Ricordo anche che è intendimento del Ministero incrementare in organico di fatto la dotazione di personale docente da utilizzare anche per soddisfare la crescente domanda del tempo pieno e del tempo prolungato richiesta dalle nostre famiglie. Tale esigenza è stata già rappresentata al Ministro dell'economia. Quanto riferito per la determinazione dell'organico del personale docente vale anche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per il quale la stessa legge finanziaria ha previsto una riduzione di 7.050 unità di personale che, sulla base di analoghi criteri valutativi, è stata definitivamente quantificata in circa 4.000 posti. Per quanto riguarda in particolare la Regione Calabria, occorre rilevare preliminarmente che dai dati in possesso, ricavabili dal sistema informativo del Ministero, nella Regione la media degli alunni per classe è pari a 18,54. Pertanto, il Ministero ha tenuto conto delle specifiche esigenze espresse dalle scuole della Regione. Vorrei anche far presente che già da alcuni anni nella Regione si sta registrando un decremento della popolazione scolastica. In particolare, per l'anno scolastico 2007-2008, era stata prevista una riduzione di oltre 5.000 allievi; invece, i dati comunicati dalle istituzioni scolastiche della Calabria, attraverso il sistema informativo, evidenziano un calo di oltre 8.000 alunni di gran lunga maggiore, quindi rispetto alle previsioni. Se il decremento fosse stato di 5.000 alunni, come previsto in un primo tempo -indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria vi sarebbe stata una riduzione di oltre 500 posti, mentre l'effettivo calo di 8.000 alunni avrebbe dovuto comportare la riduzione di 800 posti. Quindi, la riduzione prevista dal Ministero - 680 posti - è inferiore di 120 unità rispetto a quanto avrebbe dovuto essere con riferimento al solo calo degli alunni; ciò in quanto, nel determinare la consistenza degli organici delle varie Regioni - tra le quali la Calabria - si è avuto riguardo alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e di precarietà applicando indicatori e correttivi che hanno consentito di mitigare e rendere più flessibile il criterio riferito alla consistenza della popolazione scolastica. Analogamente per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la quota assegnata alla regione Calabria, quantificata sulla base della preventivata diminuzione di allievi, è stata inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata stante il maggior calo di alunni comunicato dalle scuole. Faccio anche presente che, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, l'Ufficio scolastico regionale e i dirigenti scolastici per documentate esigenze sopravvenute, potranno sempre procedere al conferimento degli incarichi che si renderanno necessari. Con riguardo, infine, al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, ricordo che recentemente è stato raggiunto l'accordo sull'atto di indirizzo generale, tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali, che è l'atto negoziale preordinato all'avvio della contrattazione di settore.

per la quale, però, non posso dichiararmi soddisfatto, perché con la sua risposta egli ha confermato le scelte di taglio operate dal Governo nell'ambito della finanziaria del 2007. evidente che ci sono problemi di contenimento della spesa, di tagli che bisogna affrontare, ma è altrettanto vero che se facciamo un'applicazione puramente burocratica dei criteri adottati su scala nazionale, non rispondiamo ai problemi e ai bisogni del territorio, delle famiglie, dei cittadini, degli insegnanti, dei lavoratori della scuola in genere. Nel corso degli ultimi sette anni, la Calabria ha già visto un taglio complessivo di circa 6.700 unità tra personale docente e personale ATA

in una situazione nella quale - come il Sottosegretario sa bene - insistono 409 Comuni, i due terzi dei quali sono Comuni di montagna, dell'interno, con collegamenti difficili e scarse possibilità per i ragazzi, soprattutto della scuola dell'obbligo, di poter accedere al sistema formativo in condizioni adeguate e soddisfacenti. La richiesta che sento di fare e di ribadire (ed era il senso dell'interrogazione, che peraltro ha preso spunto da una manifestazione promossa dai sindacati unitari della scuola e del personale non docente) è quella proprio di rivedere per il futuro questi criteri e di trovare il modo per far sì che sia possibile garantire lo stesso diritto allo studio che c'è nelle grandi città, nei nei luoghi dove ovviamente questo è più facilmente ottenibile, alle realtà rurali delle zone interne di montagna, alle piccole frazioni, evitando quindi che i ragazzi vengano di fatto privati di questa possibilità o comunque messi in condizioni di poter assolvere a questa funzione a pena di grandi sacrifici di mobilità, di spostamento, di costi per famiglie che già sono in una situazione

Vorrei segnalare, infine, un altro aspetto. Nei tagli ricadono anche quei centri territoriali per l'educazione permanente che danno una risposta immediata ai tanti lavoratori lavoratori immigrati, i quali vedono in tale strumento una possibilità di alfabetizzazione. Anch'essi sono stati sottoposti alla scure dei tagli. Mi auguro che il Governo intervenga a tale proposito.

quanti degli infortuni che si lamentano sul lavoro nel nostro Paese sono dovuti al mancato rispetto delle norme, quanti invece a insufficiente normativa e quanti ad altre cause. Ciò al fine di sapere

la richiesta è stata completamente ignorata in sede di replica da parte del rappresentante del Governo e anche da parte del relatore, ma questi evidentemente non ne aveva gli elementi, sono a chiedere una pronta risposta, considerato che a partire da mercoledì torneremo su tale argomento.